colleghi, in data 24 febbraio 2023 il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera: «Onorevole Presidente, La informo che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'onorevole Augusta Montaruli dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca. *F.to* Giorgia Meloni». Comunico che in data 24 febbraio 2023 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'istruzione

Ministro della cultura Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, di legge di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2023, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile, dimostra la sensibilità del Governo su un tema particolarmente importante, quale è quello della ricostruzione. Mi preme ricordare che già in sede di legge di bilancio, per la prima volta, abbiamo visto segnali importanti su questo tema, in quanto già nel testo approvato dal Consiglio dei ministri

ci si occupava della ricostruzione solamente nella fase emendativa della legge di bilancio. È per questo che voglio ringraziare il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro Musumeci, il commissario per la ricostruzione Guido Castelli - anche per il grande lavoro fatto in Commissione, da *trait d'union* con il Governo

quali si occupa di un aspetto fondamentale, quello della semplificazione, e reca misure volte ad accelerare e semplificare la ricostruzione pubblica nelle aree colpite dal sisma del 2009 nella Regione Abruzzo. Esso prevede che, nelle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei Comuni interessati dagli eventi sismici, si applicano le semplificazioni della disciplina dei contratti pubblici relative a interventi finanziati dal PNRR. L'articolo 2 si occupa della figura del commissario straordinario per la riparazione e la ricostruzione. Il comma 1, nella fattispecie, riguarda l'esercizio dei poteri sostitutivi in relazione agli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari per i territori colpiti dal sisma del 2016 e prevede che, laddove il Consiglio dei ministri proceda alla nomina di un commissario *ad acta*, lo debba individuare nella persona del commissario straordinario. Il comma 2 stabilisce, invece, il percorso per la nomina del commissario straordinario, che prevede sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica. Nella fattispecie - cosa molto importante all'interno di questo di questo comma - c'è anche la previsione che il commissario straordinario, entro il 31 maggio 2023, trasmetta al Governo una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione. La reputo importante perché dà la possibilità di valutare l'andamento della ricostruzione e di e di individuare, quindi, ulteriori misure per accelerare e semplificare la realizzazione degli interventi. L'articolo 3 è un'interpretazione autentica e prevede che la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso gli uffici per la per la ricostruzione, costituiti a seguito del sisma 2009, estesa al 31 dicembre 2025 nell'ultima legge di bilancio, concerne anche i titolari dei medesimi due uffici, ferma restando la durata massima dei relativi rapporti. affronta un altro argomento importante, che riprenderò quando illustrerò il lavoro della Commissione. Esso si occupa del personale degli uffici speciali della ricostruzione e proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma 2016. L'articolo 4 dispone un finanziamento di 10 milioni di euro per il 2023 del fondo regionale di protezione civile, che serve per il potenziamento del sistema regionale di protezione civile e concorre agli interventi diretti a fronteggiare le emergenze che possono essere affrontate a livello regionale senza la necessità della deliberazione dello stato di emergenza nazionale. L'articolo 5, invece, fa riferimento agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche sopprime alcune disposizioni contenute all'interno della legge di bilancio 2023, mentre l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore.

dei commissari che voglio ulteriormente ringraziare. Fondamentali per la ricostruzione sono proprio la semplificazione e la velocizzazione dei processi autorizzativi

è quella che riserva nei concorsi pubblici la percentuale del 30 per cento per orfani e coniugi delle vittime dei sismi. Come dicevo, particolare attenzione è stata data al tema del personale, che svolge un ruolo fondamentale nella ricostruzione, perché ha acquisito nel tempo tutta una serie di professionalità che rischia di essere persa con il precariato della ricostruzione. Un emendamento che è stato approvato

connesse al pagamento dell'IVA per fatture relative a interventi di ricostruzione. alla velocizzazione e alla semplificazione, tutta una serie di norme aiuta le amministrazioni a superare quei vincoli che tengono fermi

fa riferimento al personale dei Comuni dell'isola di Ischia, la quale autorizza ad assumere a tempo indeterminato il personale a tempo determinato reclutato per la ricostruzione del sisma del 21 agosto 2017. Di particolare rilievo è un altro emendamento, approvato all'interno della Commissione, che prevede delle norme per l'erogazione di risorse ai Comuni dell'isola di Ischia per compensare le minori entrate derivanti dalla sospensione dei tributi. Mi piace poi ricordare l'emendamento che va a derogare il numero minimo di alunni

dei Comuni interessati dal sisma. Da ultimo, ma non per importanza, mi piace sottolineare ed evidenziare in questa sede il rifinanziamento del fondo per i contenziosi, che che permetterà il risarcimento degli alunni che hanno subito lesioni anche gravi a seguito del crollo della scuola di San Giuliano di Puglia nel 2002.

Signor Presidente, questo decreto si può leggere probabilmente in due modi. Ci si può compiacere delle azioni esso sono state previste, sia nel testo uscito dal Consiglio dei ministri sia negli emendamenti che probabilmente verranno già presi in esame, come ci ha raccontato adesso il relatore senatore Sigismondi. Sigismondi. Fondamentalmente, si può essere contenti per l'accelerazione che questo decreto imprime, per aiutare le aree colpite da eventi sismici e calamitosi in genere. Si può essere contenti perché, chiaramente, si sveltiscono le procedure per l'affidamento dei contratti e dei lavori nelle aree citate. Siamo contenti perché questo decreto prevede la prosecuzione dei contratti di lavoro e probabilmente, se gli emendamenti verranno approvati, anche la stabilizzazione di chi lavora nel settore; il rafforzamento della struttura di missione o ancora la concessione di contributi per gli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale; nonché l'acquisizione, da parte dei Comuni,

Ma ci può essere anche un altro modo per leggere questo provvedimento. Lo si può vedere come la continuazione di un percorso, di un filo rosso che coniuga una serie di azioni. Mi voglio in particolare soffermare su quanto riguarda l'Abruzzo. Anche se sono romano, fino al 25 settembre scorso ho avuto l'onore di poter collaborare con il Presidente della Regione Abruzzo. E quindi ringrazio il mio Capogruppo e tutti i colleghi del Gruppo per avermi dato la possibilità di intervenire sull'argomento.

di due dirigenti, orgogliosamente di Fratelli d'Italia, che sono il sindaco di L'Aquila Pierluigi Biondi e il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Biondi è diventato sindaco, L'Aquila era una città morta, malgrado fossero passati otto anni dal terribile sisma: il centro era un deserto e gli operai erano gli unici esseri umani a frequentare le strade; non c'era una visione, né un programma o una strategia.

È stato per l'attaccamento alla propria terra, per la voglia di non arrendersi e la pervicace testardaggine di dare un futuro ai propri cittadini e alla propria comunità se oggi quella città e quei territori hanno ricominciato a vivere. Ecco perché questo decreto-legge si può leggere anche in è la prosecuzione di un impegno, di un Governo che fa tesoro del lavoro degli enti locali; lo sforzo diventa legge e supera ogni barriera burocratica e di carattere finanziario. Inoltre, con la norma che prevede la nomina del nuovo commissario del cratere si aggiunge un'ulteriore e preziosa tessera al *puzzle*. In questo decreto-legge c'è tutto questo.

In questo decreto, però, c'è una visione che fa la differenza e valorizza un modo particolare di chi fa politica e di chi si sente istituzione. Poi, ovviamente, vengono fuori le norme. che parla di identità, di relazione con il territorio, di sano e organico rapporto con l'ambiente. Parla di persone che hanno fatto del loro modo di far politica il buon Governo, facendolo diventare azione quotidiana e modello per tante altre città e tanti altri territori. Signor Presidente, l'Italia è purtroppo un Paese a forte rischio di calamità naturali: terremoti, alluvioni ed erosione costiera sono alcuni dei fenomeni angoscianti che si ripercuotono nel tempo. Per quanto riguarda il rischio sismico, la causa è da ricercare nella posizione geografica del nostro Paese, situato al margine di convergenza tra due grandi placche - quella africana e quella euroasiatica - spesso in movimento, dando origine a numerosi terremoti di varia entità. Alle cause naturali complesse e non facilmente prevedibili vanno aggiunte quelle antropiche, ossia gli effetti dei cambiamenti climatici, che, con un aumento della frequenza degli eventi pluviometrici molto intensi, alternati anche a lunghi periodi di siccità - come quello che abbiamo vissuto la scorsa estate e probabilmente anche in quella che ci attende comportano conseguenze abbastanza gravi: un aumento della frequenza delle frane, oppure siccità e desertificazione. L'ultimo rapporto Ispra del 2021 sul dissesto idrogeologico pone in evidenza come il 94 per cento dei Comuni italiani sia a rischio di calamità. Questi fenomeni naturali causano danni a cose e persone, danneggiano il nostro patrimonio economico e culturale (abitazioni, aziende e fabbriche) e spesso il prezzo da pagare in termini di vite umane è altissimo. Solo a L'Aquila sono morte ben 309 persone e oltre mille sono stati i feriti. Alcune città vivono in una situazione di ricostruzione perenne, nonostante gli ingenti stanziamenti statali per la ricostruzione. Tante sono le situazioni irrisolte che gravitano intorno ai terremoti italiani e tanti i danni derivanti da una cattiva politica, dalla criminalità e a volte anche dal giro di tangenti post-terremoto che rallentano la ricostruzione; senza contare i fondi che lo Stato mette a disposizione per sostenere i territori disagiati e rimborsare i cittadini dai danni subiti, che, nonostante siano sempre insufficienti e sempre in ritardo, ammontano a 120 miliardi di euro negli ultimi I danni causati dalle calamità naturali nel nostro Paese vengono drammaticamente sottovalutati e occorre agire con forza in un'ottica di prevenzione. Agevolazioni fiscali come il sismabonus e il superbonus sono fondamentali per ottenere un adeguato miglioramento sismico ed energetico del patrimonio edilizio; strumenti legislativi di questo tipo, chiari, certi e duraturi nel tempo, dovrebbero sempre essere a disposizione per favorire l'incremento della sicurezza in Italia. Il Piano proteggi Italia è stato l'unico e il più grande piano contro il dissesto del territorio per proteggere e mettere in sicurezza il nostro Paese così fragile. Nel segno della concretezza, il Governo Conte ha stanziato quasi 11 miliardi nel triennio 2019-2021, ma purtroppo è l'unico stanziamento dei Governi italiani. Ho sentito dire da molti politici scettici sui cambiamenti climatici che le future generazioni, per avere un mondo più sicuro, dovrebbero rivolgersi ai grossi Paesi che emettono gas climalteranti, come Cina, India, Stati Uniti e così via. Probabilmente è vero che senza la cooperazione di tutti i grossi Paesi non riusciremo a fermare i cambiamenti climatici. Ma proprio perché non siamo capaci di fermare la follia umana e le scelte di alcune Nazioni, dovremmo investire in resilienza, ossia nella capacità del nostro Paese di adattarsi, riorganizzarsi ed evolversi in configurazioni che migliorano la sostenibilità del sistema, lasciando un territorio meglio preparato per i futuri impatti e meno pericoloso per le future generazioni.

grazie al maggiore gettito dovuto ad IVA, Ires, Irpef e ai contributi INPS. A questo vanno aggiunti i danni evitati: logicamente, se ci sarà un terremoto, le case che hanno beneficiato del superbonus e del sismabonus non saranno da ricostruire e lo stesso vale anche per gli interventi che evitano l'acquisto di energia fossile dall'estero, che pesa nel bilancio per 40-50 miliardi l'anno. A tal proposito non si capisce perché parlamentari del centrodestra continuino a presentare emendamenti per estendere il superbonus, come l'emendamento 1.16 presentato al decreto-legge oggi in discussione, a prima firma del senatore Liris, che che chiede appunto di estendere questo famigerato superbonus fino al 31 dicembre 2025 nei territori e nei Comuni dove insistono i crateri dei sismi accaduti nel 2009 e nel 2016. fatti riproponete le nostre misure, ma con gli attacchi mediatici studiati a tavolino la coppia Giorgetti e Meloni diffonde dati non veritieri sul superbonus, frenando e intimorendo le famiglie dall'investire in sicurezza ed efficientamento energetico. Ricordo che misure come il superbonus o il sismabonus, ma anche altre come il reddito di cittadinanza, erano necessarie durante la pandemia per rilanciare il Paese, messo in ginocchio dai continui *lockdown.* E proprio grazie a queste misure l'Italia, storicamente fanalino di coda dell'Europa, è diventata la locomotiva, superando per crescita un Paese come la Germania. misure di questo tipo sono ancora oggi insufficienti e dovremmo pensare a mettere in sicurezza tutto il patrimonio edilizio italiano, coinvolgendo anche l'Europa e non litigando come state facendo per la direttiva sulle case *green.*

Le misure rivoluzionarie ideate dal MoVimento 5 Stelle ora sono state copiate anche da diversi Stati europei, mentre in Italia vengono demolite per motivi ideologici o solo perché concepite dal MoVimento 5 Stelle.

Date per scontati gli effetti dei cambiamenti climatici, che dite ci saranno, quindi non possiamo fare nulla. Ebbene, cosa propone il Governo Meloni in termini di resilienza? Cosa state facendo per mettere in sicurezza le case degli italiani da futuri alluvioni e terremoti? Cosa volete fare per evitare che la siccità distrugga il lavoro delle nostre imprese agricole e zootecniche, come è già accaduto questa estate e probabilmente accadrà sempre di più nei prossimi anni? Cosa volete fare per evitare la desertificazione dei territori?

Forse volete che i problemi della gestione delle spiagge del demanio pubblico si risolvano da sole, grazie alla vostra politica iniqua e scellerata, che non tiene conto dei rischi futuri e che probabilmente farà scomparire molti lidi e molte spiagge nei prossimi anni per l'erosione costiera?

e si sa che chi fa sbaglia. Forse voi state seguendo un'altra strategia: non fate nulla e in questo modo dimostrate di non avere idee e di non avere una visione politica e quindi vi state limitando ad obbedire a quello che i poteri forti e l'Europa vi chiedono, anche perché si tratta di un Governo - non nascondiamocelo - nato con una forte crisi di credibilità. Cosa state facendo? Assecondate l'Unione europea e i poteri forti, così vi fanno sopravvivere e governate per cinque anni? Questa è l'unica strategia di resilienza? Mi sembra una strategia poco entusiasmante. Il Il MoVimento 5 Stelle, invece, ha governato e ha avuto una visione politica nel mondo e in Europa, portando oltre 200 miliardi di euro del PNRR, risorse che in gran parte serviranno per mettere in sicurezza il nostro Paese.

cambiandole nome, probabilmente ve ne potrete intestare i meriti e questa misura potrà continuare a sopravvivere. A noi non importa se copiate le nostre idee, per noi va bene lo stesso. L'importante è permettere a questo Paese di puntare al benessere collettivo e attuare quanto prima tutte le misure necessarie e utili per poter prevenire nuovi incidenti: sicurezza, indipendenza energetica e resilienza verso l'aumento dei prezzi dell'energia nell'interesse delle generazioni future.

del decreto-legge recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile, così come avvenuto con il decreto-legge del 3 dicembre 2022, n. 186, varato dopo gli eventi alluvionali che hanno interessato l'isola di Ischia, conferma una prassi: quella di inseguire l'emergenza con provvedimenti assunti senza una visione organica e trascurando ogni forma di prevenzione. Eppure, la cura del territorio dovrebbe rappresentare una delle priorità principali, se si vuole immaginare un futuro del Paese e difendere l'incolumità e la vita stessa dei cittadini. In buona sostanza, abbiamo aspettato anche questa volta il verificarsi di un evento estremo o di una vera e propria tragedia, come quella avvenuta nelle Regioni del Centro Italia durante gli anni scorsi oppure quelle alluvionali, come nel novembre 2022 ad Ischia, devastata da frane e allagamenti, che hanno causato l'isolamento di diverse località, l'evacuazione di numerose famiglie, 1.500 sfollati e la morte di dodici persone. persone. Per quanto gli eventi di estremo maltempo, e ancor meno i terremoti, possano essere previsti, non possiamo certo dire che si tratta di eventi che dovrebbero cogliere di sorpresa né le amministrazioni locali né il Governo nazionale, almeno sul fronte fondamentale della prevenzione e dei criteri di costruzione degli edifici, dei controlli e della lotta all'abusivismo. La fragilità del territorio italiano e la sismicità dello stesso sono note e nel corso degli ultimi anni sono sono stati tanti, purtroppo, gli eventi legati al maltempo e ai terremoti che hanno sconvolto il territorio. Nessuno di questi però è stato sufficiente a realizzare un reale risveglio delle coscienze e a fare in modo che davvero si mettesse mano a una riforma organica della gestione e della manutenzione del territorio, in grado di metterlo realmente in sicurezza, insieme agli altri edifici e alle costruzioni che su di esso insistono. Un passaggio fondamentale per scongiurare tragedie o almeno per ridurre i danni davanti a eventi particolarmente violenti, garantendo per questa via la stessa incolumità dei cittadini e le reali e concrete possibilità di sviluppo turistico, è indissolubilmente legato alla salvaguardia di ambiente e territorio. In un quadro del genere e con eventi sismici che hanno devastato le nostre Regioni, mettendo in evidenza sia la fragilità del territorio sia la stessa superficialità e approssimazione con i quali si è spesso proceduto a edificare senza potenziali controlli, si è consentito anche di condonare migliaia di abusi edilizi mai sanati. Sia la tragedia di Ischia, con il conseguente decreto-legge (peraltro il Governo aveva garantito in questa stessa Aula che tale provvedimento sarebbe stato successivamente implementato), adesso la discussione su questo decreto-legge potevano e dovevano essere l'occasione per iniziare un percorso diverso, in grado di uscire dalla prospettiva inaccettabile di inseguire le emergenze, provando a tamponare ogni volta che si verifica una tragedia e mettere in campo una strategia compiuta di prevenzione e cura del territorio che avesse una visione di come cambiare passo e mettere in sicurezza il territorio delle Regioni interessate, con una visione che andasse più in là nel tempo. è al momento del tutto insufficiente e la continua bocciatura degli emendamenti che, come Gruppo Partito Democratico, abbiamo proposto in Commissione dimostra ancora una volta come il Governo non abbia la reale volontà di risolvere i problemi, lasciando inascoltati anche i numerosi appelli e le numerose richieste arrivate durante la fase delle audizioni che abbiamo svolto in Commissione ambiente. Le risorse stanziate non sono sufficienti a permettere di garantire interventi concreti, finalizzati a una reale accelerazione della ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto, con la popolazione da molti anni costretta a vivere in condizioni di precarietà ed emergenza. Proseguire lungo questa strada vuol dire dare il via libera alla prassi alla quale abbiamo assistito negli anni scorsi: una letale combinazione di mala gestione del territorio ed eventi calamitosi estremi, che si fanno sempre più frequenti e drammatici anche in relazione ai cambiamenti climatici ai quali stiamo assistendo senza aprire un dibattito franco, aperto e complessivo sul modo con cui affrontarlo. "Prevenzione" dovrebbe essere invece la parola chiave con la quale iniziare ad affrontare la questione; "prevenzione", inoltre, è anche la parola chiave che servirebbe davvero per risparmiare le risorse che si spendono in misura nettamente maggiore continuando a inseguire le emergenze piuttosto che per riparare poi i danni. Invece, nel provvedimento in esame non solo non c'è traccia di un cambio di prospettiva, ma non si rinvengono neanche le risorse necessarie a dare un contributo vero, concreto e decisivo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi calamitosi. Non solo: in maniera del tutto ingiustificata, nonostante le diverse proposte emendative presentate, si lascia fuori Ischia dagli interventi, nonostante si fosse detto, sia in Commissione che in quest'Aula, che con questo decreto avremmo recuperato le lacune del decreto Ischia; niente di tutto questo. ha deciso e ha osservato che potrebbe essere più efficace lavorare a un provvedimento *ad hoc*, preferibilmente di iniziativa parlamentare, previa audizione del Ministro competente, al fine di una non meglio precisata corretta individuazione delle coperture finanziarie, che secondo la maggioranza al momento non sono individuabili, stando ai tempi ristretti dell'esame di questo provvedimento. Sembrano - anzi, sono - tutte scuse. La realtà ci dice che continuare a rimandare non solo rappresenta un modo non efficace di governare, ma espone i territori a rischi incalcolabili, mentre non si riesce neanche a far luce e a far fronte alle calamità già avvenute, che richiederebbero un altro livello di risposte. Va sottolineato ancora una volta come le amministrazioni locali non possano essere lasciate da sole. Per questo non può essere trascurata, come si sta facendo, la necessità di sostenerle rispetto alle difficoltà esistenti nel ripagare i mutui con il MEF, a causa delle grandi difficoltà nel riprendere la regolare riscossione dei tributi. Abbiamo chiesto di aiutare le famiglie, chiedendo di non far pagare l'IMU

anche su questo punto il Governo e la maggioranza non ci hanno voluto prestare ascolto. Anzi, la bocciatura di un emendamento del Partito Democratico proprio su questo costringe i proprietari di immobili gravemente danneggiati o distrutti a pagare comunque l'imposta municipale unica, in maniera del tutto iniqua. Insomma, il Governo deve fare chiarezza e decidere se vuole aiutare o meno le comunità interessate dagli ultimi eventi calamitosi; non può certo pensare di svicolare nascondendosi dietro raccomandazioni fumose. Anche il rifinanziamento per un importo di 10 milioni del fondo della protezione civile regionale non pare adeguato alle esigenze, soprattutto se l'idea del Governo è quella di rendere efficace la gestione delle protezioni regionali senza l'attivazione dello stato di calamità nazionale: un altro aspetto che va chiarito con attenzione, soprattutto in un momento in cui, con la discussione sull'autonomia differenziata, si rischia di andare a penalizzare sotto ogni aspetto le Regioni in difficoltà. Sarebbe del tutto inaccettabile che ciò si verificasse anche davanti a emergenze che sicuramente dovrebbero essere affrontate con le stesse forze e le stesse possibilità su tutto il territorio nazionale, senza alcun tipo di differenza. Ci aspettiamo, in ogni caso, che adesso si apra una riflessione generale sulle questioni legate alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla cura del territorio e alla prevenzione del rischio sismico e in ordine alle modalità più congrue per affrontare i cambiamenti climatici in atto, cominciando dalla base e dai provvedimenti più semplici: contrastare per esempio ogni possibilità di condono e fornire alle amministrazioni locali e ai prefetti gli strumenti idonei per abbattere gli immobili abusivi.

licenziato il parere nella Commissione competente. Se si uniscono i punti del decreto Ischia, di questo decreto e di quel nuovo codice di quel nuovo codice dei contratti pubblici, dove, tra le varie criticità, ne abbiamo evidenziata una gigantesca ed enorme (quella secondo la quale nel nuovo codice si eliminerà la compatibilità geologica e idrogeologica delle opere pubbliche che saranno appaltate in Italia), ecco, se uniamo i due decreti, la mancanza di programmazione e la proposta di questo nuovo codice dei contratti pubblici, sull'altare della cosiddetta semplificazione, senza pensare alla fragilità e senza avere una tutela del territorio, il futuro per questo Paese rischia di essere peggiore e ancora più a rischio.

e fa riferimento a vicende che hanno segnato fortemente i territori che sono stati coinvolti. Da questo punto di vista, ci sono interventi importanti, sia nel testo originale, ma anche a seguito del lavoro fatto in Commissione, perché sono indubbiamente stati introdotti elementi significativi. Nel testo in esame si lavora sul tema delle gestioni commissariali, riferimento al sisma dell'Abruzzo del 2009 e di quello di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria del 2016. Sul tema della ricostruzione pubblica ci sono norme che prevedono l'accelerazione e la semplificazione delle procedure. Viene estesa la casistica rispetto a norme già previste e viene quindi consentito di proseguire e migliorare il lavoro che è stato fatto fino ad oggi. Vengono rafforzati i poteri del commissario ci sono norme anche importanti sul tema dei poteri sostitutivi. Eventuali commissari *ad acta* dovranno corrispondere alla figura del commissario straordinario: risparmiare lungaggini burocratiche ed evitare di perdere tempo, come purtroppo troppe volte è successo in passato. È importante anche il tema dell'impegno alla trasmissione di una relazione da parte del commissario, entro il 31 maggio di ogni anno,

Ci sono norme molto importanti per quanto riguarda il personale sia delle amministrazioni e dei territori coinvolti, sia degli uffici speciali, come quello per la ricostruzione di L'Aquila e quello per il cratere.

mi riferisco al fatto che si possa mantenere la presenza degli studenti, anche se non ci sono i numeri previsti dalla normativa vigente. Cito anche la riapertura dei termini per la stabilizzazione del personale e l'estensione di alcuni di questi benefici a zone che sono fuori dal cratere, ma che sono di fatto colpite da tali vicende e dal seguito delle vicende di cui parliamo. Ci sono poi il tema del rimborso IVA alle imprese e quello della riserva del 30 per cento nelle assunzioni per i parenti delle vittime.

Da questo punto di vista, ringraziamo anche chi ha svolto il ruolo di commissario, sicuramente in modo degno. Allo stesso tempo, esprimiamo anche la soddisfazione il nuovo commissario: per noi è un'espressione di soddisfazione non perché sia un collega senatore o perché appartenga al Gruppo Fratelli d'Italia, ma perché è una persona che per anni ha dedicato se stesso al tema della ricostruzione ed è stato a fianco di quelle comunità

intervenire in modo più ampio. Troviamo singolare che si metta in campo un dibattito, sicuramente importante, come quello sul cambiamento climatico, quando si parla di ricostruzione post-sismica: lo dico con un po' di perplessità.

sul tema della ricostruzione e della prevenzione, per avere norme che possano valere per il futuro, perché purtroppo lo sappiamo che questa nostra Italia è fragile

Da questo punto di vista, quindi, c'è da fare e lavoreremo anche insieme, se si riuscirà a dialogare e a non far prevalere logiche strumentali.

riunire e far tornare a vivere comunità che sono state stravolte. Nessuna nostra azione potrà restituire quei luoghi dell'anima, per citare Ignazio Silone, che così com'erano, purtroppo, resteranno confinati nell'anima e nel cuore di chi li ha vissuti. Il nostro impegno, però, per il quale devo e dobbiamo ringraziare - noi di Fratelli d'Italia - i senatori di quei territori che si sono impegnati tantissimo anche sul tema degli emendamenti per questa discussione,

a quei territori che sono la spina dorsale della nostra Italia, testimoni di resilienza e di indomabile spirito di rinascita. *(Applausi)*. Signor Presidente, gli stimati colleghi della maggioranza che ci governa ripetono spesso che ascoltano gli italiani, ma la sensazione è che facciano pedissequamente quello che gli italiani chiedono loro. Ora, vorrei ricordare che chi governa, chi stabilisce le regole che gestiranno il futuro del nostro Paese, deve perseguire l'interesse e il benessere dei cittadini non solo di oggi, ma anche di domani e dopodomani e quindi assumere talvolta decisioni impopolari, ma necessarie, per garantire tale benessere a chi ci sarà in futuro nel nostro Paese. Mi sono messo nei panni dei ragazzi che sono qui ad assistere a questa seduta e ho pensato che, se ci mettessimo a leggere il testo di questo

le disposizioni del titolo IV della parte seconda del medesimo decreto-legge recante semplificazioni e agevolazioni procedurali con maggiori poteri commissariali? Signori, questo è un provvedimento di mera burocrazia, come lo sono stati anche quelli approvati in passato. Perdonatemi, se pensavo che il vento fosse cambiato, ma non è cambiato molto. Evidentemente, si continuano a fare provvedimenti di questo tipo, demandando poi alle comunità locali, ai commissari e ai Comuni di agire. Ora, massimo rispetto ovviamente per tutti quelli che agiscono sul territorio, ma è evidente che questo sistema non funziona e che ci vorrebbe un cambio di passo.

dove ci sono versanti che potrebbero diventare pericolanti, perché la pioggia cade molto più insistente, con concentrazioni molto maggiori oggi rispetto al passato, o magari perché i terremoti possono

i manufatti che si ricostruiscono, si lavora per niente, si lavora con il rischio che la prossima volta frani di nuovo tutto, ma forse a questo non si è pensato nei ranghi della maggioranza che ci governa. Io penso che ciò sia sbagliato.

un 20 per cento, acqua di ghiacciaio e, per un 80 per cento, acqua proveniente dalle precipitazioni e dalle falde. Ma allora, se portava solo il 20 per cento, portava l'acqua dei ghiacciai; ma l'acqua dei ghiacciai non la porta in eterno, perché si stanno sciogliendo. Per cui, di questo passo, rischiamo che il Po rimanga in secca, con tutte le conseguenze del caso. Bisogna prendere provvedimenti estremamente forti, se si vuole affrontare il futuro. Non si può rimanere a nicchiare e aspettare, sperando che le cose vadano meglio. La transizione ecologica è assolutamente necessaria. Questa maggioranza ha fatto dichiarazioni pesanti contro il *green new deal*, cioè contro i provvedimenti che l'Europa ci vuole imporre relativamente al risanamento energetico degli edifici, ma ricordo che risanare energeticamente gli edifici consente di pagare bollette

quindi rischiamo di essere presi per il collo, ma almeno una proposta alternativa va fatta. Ricordo che tra i cento e i centoventi anni fa ci fu un grande cambiamento per quanto riguarda la mobilità: si passò dai cavalli alle automobili e ai treni, che si diffusero in quel periodo. Allora c'erano lavoratori che vivevano sul trasporto dei cavalli (maniscalchi, costruttori di carrozze, allevatori,

il presente disegno di legge è volto alla conversione del decreto-legge n. 3 del 2023, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. Come hanno avuto modo di ricordare i colleghi in Aula, è giusto riconoscere che c'è stata una proficua attività in sede di Commissione, che ha portato all'approvazione di diversi emendamenti presentati dalla maggioranza e dall'opposizione per migliorare il presente il presente disegno di legge. Esso contiene alcune norme che vanno positivamente nell'ottica della cura delle relazioni del territorio, però ce ne sono altre, che avrò modo di evidenziare, che sicuramente non ci soddisfano. Laddove si parla delle misure di accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite dagli eventi sismici, è normale

che andare veloce è importante, ma è più importante andare lontano. *(Applausi)*. Quando in nome della velocità, della semplificazione e dell'accelerazione si si introducono misure che rischiano di portare alcune difficoltà e non lavorare nell'ottica della trasparenza e dell'anticorruzione, soprattutto in un territorio come quello italiano, che ha conosciuto, anche nelle fasi di ricostruzione post-sisma, evidenti elementi di patologia, ci preoccupiamo. Quando invece si fa una *governance* dei poteri sostitutivi per i commissari *ad acta* e si facilita il lavoro di questi commissari e i poteri sostitutivi, siamo ovviamente favorevoli; quando si introducono misure, come quella che è stata presentata dall'emendamento a firma del senatore Sigismondi, per rassicurare i presìdi scolastici anche nelle piccole realtà interne, consentendo alle classi con un numero ridotto di alunni nelle aree del cratere sismico di evitare lo spopolamento, queste sono sicuramente disposizioni positive, che ci convincono.

il fatto di aver voluto concentrare queste misure e questi interventi soprattutto sul tema della ricostruzione del Centro Italia. Se dobbiamo muoverci, dobbiamo farlo in maniera organica, non possiamo farlo a macchia di leopardo. Tra l'altro, nel Centro Italia, visto che il criterio cronologico non si può usare, perché il terremoto dell'Abruzzo è del 2009, vorrei che ci ricordassimo anche che c'è stato un altro evento sismico che ha riguardato una Regione che conosco molto bene: quello del 2012 in Emilia-Romagna. *(Applausi)*. Credo che quello sia stato un modello virtuoso di ricostruzione post-terremoto e sono convinto che non vi siano state decisioni politiche nel voler includere o escludere altre Regioni. Se però vogliamo un presidio perché la ricostruzione venga fatta per bene, questo dipende anche dalla collaborazione che ci dev'essere delle amministrazioni locali, delle amministrazioni regionali e di tutto il sistema Italia. Il secondo punto che non mi convince è quello della protezione civile. È certo che il rifinanziamento e l'attribuzione dei fondi nel 2022-2023

il modello della Protezione civile come avanguardia del nostro Paese era costruito su una catena di comando chiara e precisa, che andava a svolgere un'attività di coordinamento interministeriale che era doveroso lasciare sotto la Presidenza del Consiglio dei ministri. Perché andate a toccare cose che hanno funzionato, cercando di costruire modelli che non sappiamo se e come funzioneranno? Ve lo ripeto: credo che quello sia stato un grave errore. Il terzo limite - come diceva anche il collega Spagnolli prima - è quello di affrontare il tema della ricostruzione, seppur nell'idea che i soccorsi e la ricostruzione debbano avvenire insieme, senza un pezzo fondamentale, che è la prevenzione. Se non investiamo nella prevenzione, non avremo mai, in un territorio come quello italiano, a rischio idrogeologico e sismico, la vera sicurezza.

È possibile che ad ogni intervento dobbiamo richiedervi quanto ancora dobbiamo aspettare, visto che ci avete chiesto voi di anticiparlo? Noi consideriamo infatti che quei provvedimenti che sono utili per il Paese (Casa Italia e Italia sicura) siano la linea della prevenzione sulla quale si fa un investimento sulla sicurezza che esce oltre la dittatura dell'emergenza.

di dare risorse alle amministrazioni locali e di aiutare i poteri di intervento, siamo favorevoli. Invece, laddove manca quello che per noi è un elemento fondamentale, cioè la visione organica dei provvedimenti che oggi adottiamo, non possiamo che continuare a muoverci nella prospettiva della riduzione del danno: è quello che faremo in questo intervento e che continueremo a fare nei prossimi interventi con senso di responsabilità e impegno civico rispetto a chi ci guarda da casa e alle popolazioni colpite dal sisma. *(Applausi)*. Faccio solo un appunto, visto che prima è stato il tema del consolidamento antisismico, che in un Paese come il nostro dovrebbe essere strutturale. Ricordo che in moltissime aree a rischio idrogeologico e sismico (parlo anche di territori del Sud, come la Sicilia e la Calabria) è inferiore al 30 per cento il numero dei Comuni che hanno adottato quello che una volta si chiamava piano regolatore generale e che oggi si chiama Come vogliamo fare prevenzione se i nostri Comuni non si dotano degli strumenti urbanistici previsti dalla legge? Andiamo verso la prevenzione per non dover rincorrere sempre purtroppo eventi catastrofici o dannosi dannosi per il nostro Paese e per la nostra popolazione.

necessari alla ricostruzione di questi territori, quindi per dare tempestività agli interventi, per accelerare e soprattutto per semplificare. lo vediamo in tanti casi, ma soprattutto in questo: la gente non crede più, è sfiduciata e quindi, se non acceleriamo e non diamo risposte

progettazioni esecutive e tutta una serie di gare e non sono stati erogati i contributi. Dobbiamo dare risposte ed ecco perché bisognava accelerare con un decreto *ad hoc* e norme specifiche.

cercando di riportare la gente nelle proprie case quanto prima. Tra le proposte, il decreto prevede l'utilizzo di crediti fiscali che siano ricondotti a meccanismi previsti per l'erogazione di contributi,

la revisione del costo parametrico su base Istat e l'ampliamento dei casi per i quali è prevista la maggiorazione del contributo concedibile, una norma quindi che stabilisca che la perdita del contributo si verifica solo dove ciò è specificatamente previsto; un pacchetto di proposte su qualificazione e su autonomia negoziale nella stipula dei contratti d'appalto, varianti, controlli, la proroga delle agevolazioni e poi l'ulteriore contributo che il decreto-legge stanzia di 10 milioni di euro per rifinanziare il fondo regionale per la protezione civile.

e i suoi componenti che, in un confronto fra maggioranza e opposizione, hanno aggiunto anche altri articoli importanti al testo che servono a dare un'accelerata, a sburocratizzare, a velocizzare, a semplificare e soprattutto a dare fiducia ai cittadini. I cittadini hanno bisogno di questa ricostruzione

Signor Presidente, colleghi, gentile rappresentante del Governo, mi ha fatto molto piacere ascoltare l'intervento del senatore Damiani, perché ero un po' perplessa sulla gestione della discussione in Aula, soprattutto per il nostro pubblico di giovani ragazzi. La partecipazione non sembrava eccezionale, invece il senatore Damiani ha ascoltato e altrettanto ho fatto io, perché è importante secondo me che ciascuna delle parti ascolti le rispettive ragioni. Andrò nella stessa direzione sulla prevenzione, perché ascoltare la parola "ricostruzione" mi suscita un senso di sconforto e di amarezza. Immagino che sia un sentimento comune in quest'Aula, perché, se si parla di ricostruzione, significa che qualcosa è andato distrutto e pare assurdo che ancora oggi, nel 2023, le calamità ci colgano di sorpresa e impreparati. Eppure, anno dopo anno, terremoto dopo terremoto, calamità dopo calamità, ci ritroviamo a contare i morti e a registrare i danni e a osservare un minuto di silenzio per le vittime innocenti, nonché a discutere di come allocare le scarse risorse dello Stato. La coperta è regolarmente troppo corta, i tempi della burocrazia troppo lunghi, e l'inefficienza dello Stato ogni volta si appalesa nella sua drammaticità. I cittadini perdono fiducia nelle istituzioni e non si riconoscono in uno Stato che appare incapace di reagire in modo adeguato ed efficace. D'altra parte, gli elementi calamitosi continuano inesorabilmente a succedersi negli anni e non si può più parlare di fatalità: ormai si deve parlare di incapacità incapacità di imparare dalle esperienze passate, di pianificare correttamente e di ammettere che il rischio naturale è la regola nel Paese delle frane, delle valanghe, delle alluvioni e dei terremoti. Non ci vuole un genio della politica per capire che prevenire costa meno che curare che agire sulle cause è meglio che porre rimedio agli effetti, ma pare che in Italia questo sia un approccio sconosciuto. Occorrerebbe essere formiche invece che cicale. Ad onor del vero, qualche formica al Governo l'abbiamo avuta: sto pensando, a proposito di prevenzione, al DPCM cosiddetto Proteggi Italia, varato dal Governo Conte I nel 2019, che stanziava quasi 11 miliardi in tre anni con l'obiettivo di mettere in sicurezza 3 milioni di nuclei familiari residenti in aree ad alta vulnerabilità, ma anche e soprattutto a mitigare il rischio e a mettere in sicurezza l'intero Paese contro il rischio idrogeologico, con la logica della prevenzione e mettendo in atto una serie di importanti misure di emergenza, prevenzione, manutenzione, ripristino, semplificazione e rafforzamento. Il MoVimento 5 Stelle, durante questi primi mesi di nuova legislatura, dalla prospettiva di una opposizione costruttiva non ha perso di vista l'importanza di insistere sulla prevenzione del rischio, nel nostro fragile territorio, per la tutela dei cittadini. Nel corso dell'*iter* di approvazione della legge di bilancio abbiamo utilizzato lo strumento dell'ordine del giorno, sottolineando la necessità di maggiori fondi per l'aggiornamento dell'inventario dei fenomeni franosi italiani che vede alcune Regioni totalmente inadempienti. Inoltre, non abbiamo perso occasione per sottolineare la necessità di stanziare i fondi necessari per il completamento e l'aggiornamento del progetto Carg

ci si è bloccati nel 1999 e nel 2020, con il Governo Conte, si è ripreso a finanziarlo. La Carta geologica dell'Italia consente di fornire dati georeferenziati utili alla corretta programmazione degli interventi per la mitigazione, la riduzione e la prevenzione. Questa Carta geologica costituisce la base per la redazione di carte tematiche derivate, in merito alla pericolosità sismica, geomorfologica, idrogeologica e geofisica, utili per la pianificazione territoriale. Ricordo inoltre che come MoVimento 5 Stelle, a prima firma del nostro collega, senatore Pietro Lorefice, è stato depositato un disegno di legge che contiene importanti disposizioni per il completamento e l'aggiornamento di questa cartografia geologica e geotematica d'Italia. Se approvato, si tradurrebbe nella disponibilità di una moderna e georeferenziata cartografia geologica, indiscutibilmente scientifico idoneo ad approfondire la conoscenza fisica e geologica del territorio. È quindi è necessario un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e di previsione, che consenta di individuare e prevedere i rischi, anziché parare i colpi. Purtroppo, nella legge di bilancio questo Governo non ha stanziato nulla per combattere e prevenire i rischi sul territorio ed è stato stanziato poco sul piano di adattamento del clima. Occorrono inoltre stanziamenti sui piani per la protezione idraulica e idrogeologica; occorre semplificare la normativa rivedere quella sul condono. Occorre una normativa sul governo del territorio, sulla rigenerazione urbana e sul consumo di suolo, perché la prevenzione dei rischi sismici e idrogeologici passa anche da un'appropriata gestione del suolo; ancora oggi abbiamo una normativa urbanistica che risale - sentite bene - al 1942. Occorre intervenire con tempestività sul meccanismo economico, che ancora favorisce l'espansione. sono capitoli di spesa che in realtà sono da leggere come capitoli di investimento. Come qualcuno diceva - qualcuno che quest'Aula apprezza sono il debito buono e il debito cattivo. Questo subito ci fa tornare alla mente un altro capitolo importante, quello relativo,

alla parte di spesa eccedente il contributo concesso per gli interventi di riparazione e ricostruzione post-sisma. Il problema è che chiaramente, avendo eliminato la cessione del credito e lo sconto in fattura, rimane solo la detrazione fiscale, che - come tutti sanno - è una cosiddetta roba da ricchi, nel senso che ci vogliono le risorse da anticipare per la misura e poi si deve avere la capienza fiscale per assorbirla. Chiaramente, in una situazione di emergenza sismica, con persone che hanno perso la casa, togliere questo sostegno per un interesse superiore sembra difficilmente comprensibile. Quindi, visto che parte della maggioranza, anche a livello locale, ha sollevato il problema dell'ingiustizia sociale che l'eliminazione di questa misura sta provocando, si auspica che essa venga reintrodotta. Concludo dicendo che la crisi climatica rappresenta la più grande sfida che l'umanità è costretta ad affrontare in questo secolo. Per essere vinta, essa necessita di un netto cambio di passo nelle politiche di mitigazione e di adattamento entro il 2030. Se vogliamo essere generosi e responsabili nei confronti delle prossime generazioni, dobbiamo smettere di essere cicale e diventare formiche, impegnandoci per lasciare i sistemi naturali e la biodiversità in uno stato migliore di quello che a nostra volta abbiamo ereditato.

danno l'impressione di non avere una visione e un orizzonte, anche su temi delicatissimi come quello in esame. In generale, che altro deve accadere in questo Paese, tra siccità e bombe d'acqua, tra dissesto idrogeologico e scioglimento dei ghiacciai, per comprendere che la lotta ai cambiamenti climatici e l'impegno per una sostenibilità produttiva di modi di produrre, di vivere, di muoversi e di consumare sono un imperativo per tutti? Che altro deve accadere per comprendere che immediati e risolutivi interventi per il riassetto e il rammendo del territorio sono fondamentali per il futuro del Paese e per la prevenzione di tragedie e calamità? Di solo presentismo, anche in questi campi, si muore. A proposito di queste calamità, rappresentano per noi una tappa fondamentale - ma crediamo la - la definizione e l'approvazione di un serio codice della ricostruzione, che possa aiutare l'Italia ad avere modelli seri e flessibili, validi per diverse circostanze. Il provvedimento in esame si colloca in un quadro nel quale molti cittadini, che comunque avevano dato fiducia a questo Governo e a questa maggioranza con il voto, voto, manifestano contrarietà per le discrepanze tra gli annunci fatti in campagna elettorale e i provvedimenti concretamente adottati, sui quali lo voglio far rilevare - si sono già consumate nove richieste di fiducia. Ripeto: nove, tre al mese. Se - come dite - volete durare cinque anni, ne dovrete porre quasi 180. Del resto eravate pronti, e si vede. A porre le questioni di fiducia eravate prontissimi! Devo dire che è una pratica usata un po' da tutti i Governi, di centro, di destra e di sinistra.

non sono state date quelle risposte strutturali, che pure necessitavano e di cui il Paese aveva bisogno. Anzi, secondo noi sono state date zero risposte alle questioni vere, legate alla crisi energetica, al sostegno alle imprese e alle famiglie, alla sanità pubblica, ai salari, agli stipendi erosi dall'inflazione, al fatto che l'Italia ha i salari tra i più bassi d'Europa, e potremmo continuare. Quello che vediamo, poi, è anche una certa miopia. Magari per cercare di gratificare alcune categorie avete persino rischiato e state rischiando di rompere i rapporti con l'Europa: pensiamo a quello che sta succedendo con la vicenda dei balneari, al richiamo del presidente Mattarella e al rischio della procedura di infrazione da parte dell'Europa.

Sappiamo anche noi che la misura del superbonus, così come era concepita e attuata, presentava delle criticità per i conti pubblici, pur avendo dato un importante scossone al settore dell'edilizia e all'indotto. Era chiaro che si dovesse costruire una modifica delle norme, ma modo e sostanza con i quali avete agito sono improvvisati e ingiusti. Avete detto che era questa anche la vostra intenzione, che si trattava di trovare i giusti equilibri, ma non è così. Avete fatto un *blitz* e tantissime imprese e famiglie che aspettavano giuste decisioni si sono ritrovate veramente in una situazione di drammatica difficoltà. Avete bocciato anche i nostri emendamenti

con lo Stato e le regole, ma favorite chi non li rispetta, come è avvenuto con gli evasori fiscali, con i no vax e via condonando. Ecco perché è intollerabile questo atteggiamento. Nel merito, sono a grave rischio di blocco parti importanti del piano di ricostruzione, a seguito degli abbattimenti degli edifici che sono in corso, anche in virtù degli incentivi programmati. tratta di una situazione delicata. Voglio dare atto al commissario Castelli di aver raccolto questo nostro appello, che peraltro era anche l'appello di tanti sindaci e di tante forze sociali di tutti i territori del cratere. il commissario Castelli sabato, a Norcia, in un'occasione di fiducia e di speranza, per l'accensione della fiaccola di San Benedetto, in una bella manifestazione sui prodotti tipici locali. Anche in quella sede il commissario ha rafforzato questo impegno. Ora però, al di là della volontà espressa dal commissario, chiediamo al Governo di fare sul serio, di non limitarsi a fare promesse e di intervenire perché la misura del superbonus venga corretta come è necessario fare - e soprattutto venga ripristinata per le zone terremotate, perché altrimenti sarebbe un'ingiustizia sopra un'altra ingiustizia. Infine, avete manifestato immotivata chiusura anche su tanti emendamenti del Partito Democratico e sui riconoscimenti risarcitori ai parenti delle vittime.

insoddisfazione anche per la bocciatura degli emendamenti finalizzati all'assunzione di personale per i parchi, garantendo loro stabilità, al supporto psicologico e al patrocinio legale gratuito alle vittime dei disastri, per le risorse da destinare alla lotta ai mutamenti climatici nell'ambito del fondo per la protezione civile. Sono state bocciate anche le nostre proposte dedicate all'alluvione di Ischia, sulla sospensione fiscale, sulle misure per rafforzare gli organici, su quelle relative al trasporto scolastico. Vediamo silenzi imbarazzati dei parlamentari di maggioranza che nei territori rilevano la situazione, ma poi qui sono costretti a votare un provvedimento che essi stessi condividono poco. Insomma - concludo Presidente - nelle aree della ricostruzione è capitato, è capitato, e non solo a me naturalmente, di toccare con mano dolore, angoscia per le morti, le tragedie, le case crollate, per i rischi di spopolamento e desertificazione di alcuni tra i territori più belli del nostro Paese, la fascia appenninica, l'Italia di mezzo. Ma a quel dolore, a quella tragedia hanno fatto poi seguito, grazie all'impegno dei Governi e delle Aule parlamentari, fondi per la ricostruzione e altre iniziative. Non ci siamo voltati dall'altra parte, e questo è vero. E io do atto anche al lavoro dei precedenti commissari, a partire dall'ultimo. Un ringraziamento voglio rivolgere anche in questa sede a Giovanni Legnini, che ha velocizzato con le sue ordinanze la ricostruzione che oggi è un qualcosa di più di una speranza, un qualcosa che si avvia ad essere concreto. Occorre rafforzare però quella fiducia, non tradirla con provvedimenti sbagliati. Occorre lavorare per accelerare, e non per demolire, quella speranza con questi provvedimenti discutibili e dare forza con due parole chiave: unità e coesione. Per noi sono parole chiave, che però purtroppo sembrano mancare visibilmente a questo Governo e alla sua maggioranza.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, mi pare che Stefano D'Arrigo, lo scrittore siciliano, abbia detto che in Italia ci sono due grandi categorie di persone che si occupano di politica, due partiti: uno è il partito del visto con gli occhi, l'altro è il partito del sentito dire. Io sul tema sisma sono d'ufficio iscritto al partito del visto con gli occhi, visto che ore 3,36 del 24 agosto del 2016 ero sindaco. Successivamente, finito di fare il sindaco, ho fatto l'assessore alla ricostruzione e ora mi trovo a fare il commissario straordinario. con l'attenzione che da sempre riservo al tema del sisma 2016, che questo è un buon provvedimento. questo è un buon provvedimento. E invito davvero anche le opposizioni a valutare l'opportunità di votarlo, perché sarebbe non solo un bel segnale, ma anche una restituzione importante e significativa ai molti sindaci, ai molti governatori e a coloro i quali, affollando quella che io definisco la comunità del sisma, chiedevano provvedimenti

Quindi, dobbiamo guardare a questo provvedimento come a un intervento che probabilmente doveva e poteva essere fatto prima e che va a correggere, almeno per quanto riguarda il sisma 2016, alcune distorsioni che rischiavano di compromettere la ricostruzione stessa, la sua tempestività, la sua adeguatezza. Cito, fra le diverse cose, tre questioni che sono nodali, quale che sia poi il proprio partito (quello del Innanzitutto, cito l'assoluta necessità che la ricostruzione possa disporre di un *set* di professionisti della pubblica amministrazione che possano essere stabilizzati, in maniera tale che quegli operatori pubblici possano, nel tempo, consolidare la propria funzione decisiva.

proposto di tenere in considerazione? Il fatto che - come è noto - i nostri ragazzi, quelli che lavorano nei Comuni, se non hanno una prospettiva, se ne vanno. Non ci lavorano a Pieve Torina, non ci lavorano a Servigliano; ci lavorano per un po' e poi se ne vanno e grande è la concorrenza, anche da parte del privato. Abbiamo una assoluta necessità, quindi, non solo di consolidare l'apparato amministrativo di quei Comuni (sono 138), ma anche di consentire a quegli stessi Comuni, Comuni, esaurita la ricostruzione, di mantenere dei presidi, che necessariamente devono disporre di una pubblica amministrazione adeguata. Il tema della stabilizzazione del nostro personale

la formazione delle stesse classi; ed è più complicato da mantenerle nella misura in cui si affidano quelle scelte agli *standard* numerici che sono quelli nazionali e generali. La chiusura delle classi e il rischio di spopolamento, indotto proprio dalla perdita del servizio dei servizi, che lega in maniera più significativa la scelta delle famiglie alla decisione di rimanere in quei posti, oggi possiamo dire superati nella misura in cui, fino all'anno scolastico 2028-2029, si potrà derogare a quelli che sono gli *standard* numerici per la formazione di classi, che quindi potranno essere mantenute. Certo: ciò non esclude che bisognerà essere intelligenti e ragionevoli e cercare comunque di contrastare fenomeni di spopolamento di classi troppo poco nutrite di studenti. però, ci chiedevano da anni e questo siamo riusciti a fare. Non è un intervento puntuale nel senso deteriore del termine, ma è intervento necessario, che arriva, e speriamo di poter dire non tardivamente, ma che doveva arrivare. Ce ne sono altre di tali questioni, ma non voglio attardarmi su questi aspetti. Non so quanti di voi conoscono quanto accaduto a coloro i quali hanno perso la propria attività produttiva, che l'hanno vista lesionata dal sisma, da una furia che - non lo dimentichiamo - in quella sequenza fatta

ancora oggi devono anticipare l'IVA sulla lavorazione dei materiali. Ma vi rendete conto? L'albergatore di Ussita, posto meraviglioso, luogo delle mie amate Marche, che non lavora da anni, deve anticipare l'IVA sulla ricostruzione. Queste non sono cose da considerare parte di una valutazione ideologica o partitica o delle considerazioni che stiamo mettendo in campo: sono necessità assolute che il Governo ha voluto sostenere anche con delle risorse, fondamentali per fare in modo che queste legittime aspirazioni fossero poi suffragate. Sono scelte politiche, che io credo sarebbe bene, giusto e auspicabile potessero essere condivise, proprio perché accedono a quei dettagli in cui - come è noto in cui - come è noto - si annida il diavolo e che, spesso e volentieri, non consentono le giuste e necessarie azioni, che sono complesse e tanto tanto più complicate. Veniva ricordato prima il sisma del 2012 dell'Emilia-Romagna. Ripeto ancora una volta che non si devono fare gerarchie, perché ogni tragedia ha una sua storia. È evidente, però, che la caratteristica precipua del sisma del 2016 è che si è scaricato in un'area appenninica Anche fare cantieri è complicato e significative della nostra Nazione, rispetto alla quale - è un altro argomento che voglio sottoporre all'attenzione di chi magari ancora non ha deciso di votare favorevolmente questo decreto-legge

sofferenti per una gelata demografica ingravescente anche prima del 2016. Rispetto a quest'ultimo tema, che è la seconda gamba della ricostruzione, noi ambiamo a dire e vogliamo farlo, sapendo quanto sarà anche complesso - che, oltre alla ricostruzione, è necessario provvedere alla rigenerazione e alla rivitalizzazione economica e sociale Sono state fatte delle cose; io ero parte della cabina di coordinamento, insieme al commissario Legnini, che anch'io ringrazio per quello che ha fatto. E devo dire che abbiamo già cominciato a lavorare in maniera tale che la seconda gamba della ricostruzione, ovvero la rivitalizzazione, sia sempre presente nell'agenda del commissario, dei

dobbiamo curare, perché siamo in una fase che ancora richiede molta attenzione sull'attuazione concreta delle molte risorse assegnate, che ora devono essere messe a terra e impiegate con scrupolo. questo decreto-legge attribuisce al commissario anche il ruolo di curare la riparazione, il rammendo, la riconfigurazione di un flusso minimo vitale che sappiamo essere ancora possibile recuperare, a un'azione già promossa nel fondo complementare area sisma, che ha consentito anche di stimolare economicamente quelle aree. Il commissario che si occupa di riparazione e di ricostruzione è colui il quale, insieme alle Regioni e ai Comuni, in una logica multilivello, potrebbe arrivare a far sì che la ricostruzione del terremoto del 2016 possa diventare un modello per le altre aree interne. Guardate che dalle nostre parti -lo dico perché sono di quelle zone - abbiamo avuto solo la sventura di vedere anticipato l'esito di una crisi delle aree interne che da tempo

com'era e soprattutto come sarà, tenendo conto che il patrimonio edilizio deve avere quelle caratteristiche e quegli *standard* che prefigurano luoghi in cui sarà possibile tornare a vivere, anche perché è certo che vi siano connessione, sicurezza, solidità sociale e soprattutto capacità di intercettare intercettare la modernità. Una parte consistente della nostra tradizione nazionale ed europea nasce da quelle parti: noi siamo convinti che, tra le tante cose possibili, sarà possibile continuare questo questo percorso, sapendo che la rinascita dell'Italia centrale è di per sé anche la ricostituzione del cuore della nostra Italia.

è naufragato davanti alle coste crotonesi. Il bilancio ufficiale è drammatico e registra al momento 64 vittime, di cui 14 minori, ma il numero potrebbe essere molto più alto. Le immagini che tutti noi abbiamo visto sono veramente drammatiche. Ci troviamo di fronte a una tragedia che non può lasciare nessuno indifferente. Lo ripeto: nessuno. Consentitemi di rivolgere innanzitutto il mio ringraziamento a quest'Assemblea per l'attenzione che dà ai tanti operatori, agli uomini e alle donne in divisa, ai tanti volontari che sono tuttora impegnati in difficili operazioni di soccorso. Nessuno ci ridarà indietro quelle donne, quei bambini e quegli uomini. Niente e nessuno potrà sicuramente lenire il dolore dei loro familiari, ma di sicuro possiamo, anzi dobbiamo fare in modo che questi eventi non si ripetano. Perlomeno dobbiamo seriamente provarci. Tutti - come ha ricordato autorevolmente il Presidente della Repubblica - a partire innanzitutto dall'Europa, abbiamo l'obbligo anche morale di impegnarci maggiormente, affinché quello che abbiamo visto a Steccato di Cutro non si ripeta in futuro.

è noto, domenica scorsa in Italia si sono svolte le elezioni primarie del Partito Democratico; oltre un milione di persone si sono recate ai seggi ed è stato uno straordinario esercizio di democrazia che è valso e ha un valore anche al di là del Partito Democratico stesso. Tutte le forze politiche, infatti, quando c'è un esercizio di democrazia devono farne tesoro e attribuirgli un valore importante. Purtroppo in quella giornata, in quello straordinario esercizio di democrazia, proprio mentre svolgeva le sue funzioni di scrutatore è venuto a mancare Daniele Nocera, che era un iscritto al Partito Democratico, un ingegnere, un amico. Tenace

una moglie e una figlia di due anni. Accanto a lui ci stringiamo come Gruppo Partito Democratico, come comunità democratica, ma sono convinto che lo faremo anche attraverso il ricordo, il saluto e l'abbraccio di tutta l'Assemblea del Senato. il mio intervento è un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché protegga tutti i bambini che vivono nei siti inquinati, tra cui quello di Taranto. Pochi giorni fa è stato pubblicato, a cura dell'Istituto superiore di sanità, il sesto Studio Sentieri sullo stato di salute delle popolazioni che vivono nei siti inquinati italiani di interesse nazionale. Lo Studio Sentieri ha dedicato particolare attenzione allo stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto, documentando nel periodo 2013-2017 un eccesso di malformazioni congenite, ricoveri per tumori maligni, tumori del sistema nervoso, nonché un eccesso di leucemie e decessi. Quei bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti funzionavano e gli impianti funzionano ancora, seppur sotto sequestro della magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione. Allora, nel lontano 2012, si consentì la prosecuzione dell'attività produttiva perché si ritenne che le nuove prescrizioni e le nuove tecnologie fossero tali da bilanciare le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita. La morte e la malattia dei bambini tarantini devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata. Il recente decreto impianti di interesse strategico nazionale ripropone, tra le altre cose, oltre allo scudo penale, lo stesso generico e fallace criterio del bilanciamento, per validare modelli organizzativi atti a prevenire reati e consentire ancora la prosecuzione dell'attività produttiva dell'impianto siderurgico di Taranto. Non sta a noi dirle, Presidente, quale sia la cosa giusta da fare quando le verrà chiesto di apporre la sua firma in calce a quel decreto-legge, che non condividiamo. Le chiediamo semplicemente di considerare di interesse strategico nazionale la vita dei bambini dell'intera Nazione, che vive il triste e gelido inverno della denatalità; di tutti i bambini che vivono nei SIN italiani e in particolare dei bambini di Taranto, città che recentemente l'ONU ha incluso tra le zone di sacrificio, zone che - come affermato dalla stessa Organizzazione internazionale - rappresentano la peggiore negligenza immaginabile dell'obbligo di uno Stato di rispettare, proteggere e realizzare il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile. Chiediamo a lei, presidente Mattarella, di proteggere e garantire tutti i nostri bambini, futuro pulsante della Nazione. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questo pomeriggio, ha stabilito di integrare l'ordine del giorno di domani con l'esame della sede redigente del disegno di legge istitutivo di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, già approvato dalla Camera dei deputati, e di rinviare alla prossima settimana le votazioni per i componenti dei consigli di presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria. Gli emendamenti al decreto-legge sulla ricostruzione a seguito di eventi calamitosi dovranno essere presentati entro le ore 19 di oggi. Gli emendamenti al disegno di legge recante modifiche alle disposizioni per il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali devono essere presentati entro le ore 13 di domani.

e connessi - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie